Onorevoli colleghi, è presente in tribuna una delegazione dell'Assemblea nazionale della Repubblica del Vietnam, alla quale inviamo un nostro caloroso saluto.

recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

credo che la replica debba toccare alcuni argomenti che sono stati evidenziati in sede di discussione generale

il G8, la discontinuità nella cessione di rami d'azienda e di società in amministrazione straordinaria e l'interpretazione autentica legata al *décalage* del

non ho trovato pertinenti alcune valutazioni sugli emendamenti presentati da colleghi e che pure sono stati esaminati e magari anche respinti dalla Commissione, nel metodo con cui ha affrontato profilo rigoroso di valutazione degli emendamenti in ordine ai pareri espressi dalla Commissione bilancio, alcuni dei quali sono intervenuti - li esamineremo oggi in Aula - successivamente al termine dei

la proposta dei senatori Zanetta, Grillo ed altri non soltanto conteneva una riduzione sostanziale dei compensi degli arbitri del 50 per conteneva la vera norma di moralizzazione nel solco in cui si è andati negli ultimi anni, e cioè la assoggettabilità del giudizio arbitrale, la riconduzione del tema arbitrale nell'ambito di un procedimento civile accelerato. Sono emersi, nel corso del dibattito, alcuni elementi rilevantissimi che pure sono stati evidenziati in sede di

quanto è emerso nel corso delle audizioni e cioè il verificarsi, durante la costruzione della Salerno-Reggio Calabria, di gravissimi atti di illegalità. In particolare, tra i più gravi, quello di frode di identità dei lavoratori, particolarmente delle imprese subappaltatrici il fatto, denunciato dalle organizzazione sindacali, che in moltissimi casi vi sono buste paga assolutamente regolari e contributi regolarmente versati, ma corrispettivi pagati agli operai nell'ordine di 30 euro giornalieri per gli operai comuni e di 45 euro giornalieri per gli operai specializzati. È un fatto intollerabile, che quest'Aula deve

chiederemo al Governo di intervenire in maniera che la Salerno-Reggio Calabria diventi un corridoio di legalità. Rubo la frase al collega Ranucci perché descrive perfettamente quello che il Governo dovrebbe fare - e che, a mio parere, tutto il Parlamento deve chiedere all'Esecutivo - sulla Salerno-Reggio Calabria, anche adottando misure di natura straordinaria.

quell'area ad evolversi anche dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista civile. Evitiamo di imbarbarire ancora di più i rapporti e facciamo emergere situazioni che certamente non vanno premiate.

che assumeremo oggi - mi rivolgo anche alla senatrice Fioroni - preveda che anche gli enti pubblici siano interessati da una restituzione

nel 1962 producevano in proprio l'energia, in quanto ne consumavano in grandi quantità, e che nel percorso di nazionalizzazione hanno visto

Credo sia giunto il momento in cui si debba tornare a parlare in Conferenza dei Capigruppo di questa esigenza. Penso che il senso di responsabilità di tutti i Capigruppo e dei singoli senatori ci dovrebbe portare a regole di comportamento condivise, per il rispetto del ruolo che svolgiamo. Prego, senatore Cicolani,

di produrre una discontinuità anche nei rapporti di lavoro tra la situazione precedente e quella di arrivo. Mi sembra

ha causato una perdita di prodotto interno lordo e ci priva oggi di risorse importanti per riavviare lo sviluppo. L'emergenza prezzi degli ultimi 18 mesi rischiava di bloccare i lavori in corso nelle infrastrutture,

L'urgenza del provvedimento è quindi chiara ed è stata confermata, oltre che dagli interventi dei senatori Gallo e Zanetta, anche da quelli dei senatori dell'opposizione Marco Filippi, Ranucci, De Castro e Fioroni che, facendo riferimento

Do atto quindi ai senatori Legnini, Morando e Azzollini dei significativi rilievi di carattere metodologico sollevati, ed esprimo gli orientamenti della Presidenza al riguardo. Per quanto riguarda la questione di proponibilità, riconosco al Presidente dell'8ª Commissione di aver valutato gli emendamenti presentati e successivamente approvati in quella sede secondo criteri conformi ad una prassi consolidata. Alla luce di tale prassi va considerata anche l'assenza di precedenti che vedano la Presidenza dichiarare improponibili emendamenti approvati dalla Commissione di merito a disegni di legge di conversione di decreti-legge. Pertanto ritengo non vi siano oggi le condizioni per pronunciare la improponibilità degli emendamenti della Commissione né di alcun altro emendamento presentato al provvedimento in esame. Ciò anche alla luce della considerazione che, non consentendo la prassi attuale di dichiarare inammissibili emendamenti già dichiarati ammissibili e accolti in Commissione, si verrebbe a creare una incomprensibile difformità fra tali emendamenti e quelli successivamente presentati in Assemblea da parlamentari sia dell'opposizione che della maggioranza. Gli emendamenti presentati hanno tuttavia quantomeno aspetti di attinenza al contenuto del decreto-legge. Una diversa decisione della Presidenza assumerebbe poi - tenuto conto della prassi più volte richiamata - un valore in un certo senso retroattivo riflettendosi sulle deliberazioni già assunte dalla Commissione. Pertanto, allo stato degli atti, essa non può venire adottata. Per il futuro dei nostri lavori, con particolare riferimento alla sessione di bilancio, esprimo qui - e lo farò formalmente nei prossimi giorni una forte raccomandazione ai Presidenti delle Commissioni in ordine ad un puntuale vaglio di ammissibilità degli emendamenti a decreti-legge anche sotto il profilo richiamato dalla recente giurisprudenza costituzionale circa la necessaria coerenza per materia con il testo. La Presidenza si riserva fin d'ora di valutare tali emendamenti con l'opportuno rigore, e di dichiararne se del caso l'improponibilità qualunque sia la loro provenienza, dunque anche se approvati in Commissione o proposti dal Governo. Quanto poi ai profili finanziari - richiamati con acutezza dai senatori Morando ed Azzollini - esprimo un invito al Presidente della Commissione bilancio per un vaglio rigoroso e puntuale delle conseguenze finanziarie dei testi e degli emendamenti in discussione, avvalendosi il più possibile dell'ausilio informativo del Governo, al quale rivolgo il medesimo invito ad esprimere la più fattiva collaborazione con la Commissione bilancio. In particolare, a parte la conseguenza procedurale in termini di improcedibilità per gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio abbia già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, rivolgo un appello al Governo affinché valuti se presentare, all'inizio della sessione di bilancio in Senato, un emendamento che allinei le tabelle del disegno di legge finanziaria con lo stato della legislazione vigente, in maniera da permettere al Senato stesso di esaminare testi improntati al criterio della veridicità. Invito altresì il Governo ad informare con la maggiore tempestività possibile la sede propria della 5a Commissione, durante l'esame dei documenti di bilancio, circa lo stato degli emendamenti presentati ai vari provvedimenti in discussione. Ciò nel caso in cui gli emendamenti, avendo conseguenze finanziarie, vadano ad incidere direttamente sui documenti di bilancio e in particolare sul disegno di legge finanziaria. Il Governo infatti è a perfetta conoscenza anche dell'*iter* dei provvedimenti presso la Camera dei deputati. Il risultato di tale collaborazione dovrebbe ugualmente essere

*(PD)*. Signor Presidente, mi riferisco alla seconda parte della sua comunicazione, quella relativa alla questione che ho cercato di sollevare ieri nel corso della nostra discussione. Non vi è dubbio che l'ipotesi da lei avanzata, cioè che all'inizio dei lavori della Commissione bilancio, e in generale del Senato, sulla legge finanziaria e sulla legge di bilancio il Governo si faccia carico di presentare un emendamento alla legge finanziaria stessa (qualora si tratti di tabelle) o alla legge di bilancio, per fare in modo che in partenza il disegno di legge all'esame della Commissione bilancio abbia recepito le conseguenze dell'approvazione di testi di legge che incidono, ad esempio, sulle tabelle (come ieri ho cercato di richiamare),

fare una verifica delle nostre procedure di decisione di bilancio a tale propositoanche nella Giunta per il Regolamento per verificare se l'apporto di qualche piccola correzione possa aiutareil Senato In ogni caso, per questo aspetto, credo che la sua comunicazione possa fornire sia alla 5a Commissione permanente che al Governo indicazioni utili per una migliore gestione della difficile fase che si è aperta con la la sessione di bilancio e la contemporanea discussione di provvedimenti di legge onerosi che si collocano all'interno della conversione di decreti-legge.

La ringrazio, senatore Morando, anche per avere posto all'attenzione della Presidenza un problema che, secondo il sottoscritto, assume una rilevanza strategica nella gestione dei lavori dell'Assemblea durante la sessione di bilancio.

i rilievi regolamentari e costituzionali che abbiamo proposto ieri. Apprezziamo lo sforzo che lei ha compiuto. Tuttavia, relativamente alla prima parte della sua decisione, quella cioè che attiene all'improponibilità degli emendamenti estranei all'oggetto del contenuto del decreto-legge in fase di conversione, dobbiamo evidenziare una non condivisione. Lei ha assunto

in cui è corrente, è certamente contraria ai precetti costituzionali a cui mi sono riferito nella giornata di ieri, in particolare all'articolo 77 della Costituzione, nonché a a norme regolamentari precise che vigono, come ho detto ieri, in questo e ancor di più nell'altro ramo del Parlamento e che sono state oggetto di censure precise da parte della Corte costituzionale e della Presidenza della Repubblica. Lei ci insegna che la prassi, pur costituendo indiscutibilmente una fonte indiscutibilmente una fonte regolamentare per i nostri lavori, giammai può porsi in contrasto palese e aperto con le norme ed i principi costituzionali. Credo che lei abbia abbia condiviso l'impostazione complessiva del rilievo che abbiamo formulato sul punto, laddove mi sembra faccia trasparire, con la sottolineatura dell'oggi sul testo, che per il futuro intenderà invitare espressamente i Presidenti delle Commissioni (e comunque l'Assemblea) Lo faremo in via ufficiale, senatore.

al secondo punto si è già pronunciato il collega Morando, quindi faccio solo rilevare che il Governo in più occasioni è stato chiamato a fornire chiarimenti e informazioni sulle appostazioni di bilancio, sui rilievi di carattere finanziario che la Commissione ha man mano sollevato, ma non sempre mostra una puntualità informativa; anzi, la inviterei a Per questa ragione le chiedo, signor Presidente, di investire della questione la Giunta per il Regolamento che, come ci è noto, ha poteri precisi in relazione alle questioni interpretative e regolamentari da noi proposte, che assumono un rilievo molto significativo proprio in considerazione delle affermazioni che lei ha fatto con la decisione comunicataci questa mattina. Le chiederei, signor Presidente, sia relativamente all'approfondimento delle questioni che lei ha posto che lei ha posto ed in parte risolto, sia soprattutto per le tematiche che riguardano i comportamenti futuri, di investire subito della problematica la Giunta per il Regolamento e, comunque, di farlo in tempi ragionevolmente brevi.

chiaramente improponibili e poi ad investire della questione la Giunta per il Regolamento, allora si può anche attendere qualche ora e qualche giorno per investire della questione la Giunta stessa; altrimenti ritengo che, proprio per poter meglio vagliare, approfondire e determinarsi sui punti che lei ha evidenziato, sarebbe necessario riunire subito la Giunta per il Regolamento.

le istanze che ieri sia io che i senatori Morando e Legnini le avevamo posto. Quindi personalmente sono profondamente soddisfatto delle sue dichiarazioni e del modo in cui

ha detto, perché in questo provvedimento i problemi di estraneità di materia sono francamente molto circoscritti dato che l'ampiezza stessa dei campi in cui questo provvedimento *ab origine* interviene ha consentito una emendabilità che sul piano della materia è abbastanza coerente con l'impostazione; dico "abbastanza" perché non è completamente coerente, però già su questo provvedimento i problemi francamente non ci sono stati per la materia. È chiaro che per il futuro, e con riferimento ad altri provvedimenti, il suo richiamo alla modifica della prassi che intende determinare a partire dal prossimo provvedimento secondo me è soddisfacente perché avvicina i lavori di quest'Aula sempre più al dettato costituzionale e alla giurisprudenza costituzionale. Per quanto riguarda invece i profili finanziari, signor Presidente, che hanno investito più pertinentemente questo provvedimento, ma anche altri, naturalmente, accolgo con soddisfazione l'invito da parte sua al rigore estremo. Le assicuro che già per questo provvedimento la Commissione nel suo complesso (ringrazio per questo i colleghi dell'opposizione che nella nostra Commissione danno un contributo essenziale e costruttivo

con rigore, così come abbiamo fatto, ma anche con maggior rigore aderendo alla sua ispirazione. Signor Presidente, apprezziamo soprattutto quel richiamo alla definizione delle grandi tabelle - della tabella C in particolare - che sono l'oggetto dei cosiddetti tagli lineari e che potrebbero compromettere l'operatività. Mi pare che la soluzione da lei scelta, il riallineamento di quella tabella all'inizio dell'esame della legge finanziaria, ci consentirà un miglior lavoro. È chiaro che, dell'esame di questi decreti-legge, dopo il riallineamento della tabella all'inizio della sessione di bilancio, sarà nostra cura valutare con estremo rigore. Altrettanto opportuno è il suo richiamo ad uno sforzo anche bicamerale, perché una parte degli emendamenti è presentata nell'altro ramo del Parlamento, e credo che la sua

l'illustrazione da parte del Governo di una puntuale ricognizione dei prelievi fatti dal FAS e dei coefficienti utilizzati per capire quanto era stato già attinto, talvolta forse impropriamente, dallo stesso Fondo. Per fortuna comincia la sessione di bilancio nella quale la legge finanziaria, con un emendamento della Camera, della Camera, ridetermina la quota dei fondi FAS da dare direttamente alle aree sottoutilizzate nella misura minima dell'85 per cento. In quella sede sarà cura della Commissione bilancio fornire alla Commissione, prima, e all'Aula, poi, un'esauriente relazione su ciò che accaduto. Mi pare, aderendo anche al senso generale della sua impostazione, di poter fare di quel Fondo, particolarmente ampio e delicato,

compostamente soddisfatta del dibattito intervenuto questa mattina e auspica che le risposte che ha dato all'Aula possano

Sugli aspetti finanziari ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Morando, che ha preso atto dello sforzo della Presidenza di porre in essere nuove regole che che inseriscano procedure di più preciso allineamento tra le previsioni contenute nelle tabelle della finanziaria e gli interventi *in itinere* che attingono alla finanziaria determinandone un cambiamento delle linee.

è estremamente sensibile alle alte professionalità di esponenti sia di maggioranza che di opposizione su questi temi; non foss'altro perché sia la maggioranza che l'opposizione

Sostanzialmente, da ora in poi, anche se un emendamento dovesse essere ritenuto ammissibile dal Presidente di Commissione, la Presidenza stessa dell'Aula si riserva la facoltà facoltà di renderlo improponibile; lo farà però da domani in poi, perché innova una prassi e lei mi insegna che quando si innovano le prassi è giusto darsi un momento di verifica, un momento di verifica, di stasi per informare tutti che da domani le regole cambiano, proprio perché, essendo prassi e non regole scritte, non essendo fonte giuridica autonoma, ma soltanto consolidata e derivante dalla consuetudine, occorre un momento di decantazione e di informazione nei confronti dei soggetti chiamati poi ad applicare queste regole non scritte.

di un sostanziale emendamento del Governo stesso su una consistente utilizzazione dei fondi FAS. Quindi, la Giunta per il Regolamento verrà chiamata senz'altro ad affrontare questo tema in occasione delle prossime riunioni.

l'innovazione alla prassi dalle prossime sedute e non da questa. Se dovessi accedere alla sua richiesta sin da adesso nel modo e nei termini che lei ha posto, sostanzialmente eluderemmo la volontà di modificare la prassi da domani ma l'attueremmo immediatamente; non mi sembrerebbe conducente.

Vorrei che sia chiaro - ma lo è da quanto lei ha detto - che, per i prossimi decreti-legge, i Presidenti di Commissione, prima, e poi eventualmente la Presidenza del Senato dichiareranno inammissibili gli emendamenti estranei agli oggetti dei decreti stessi. Naturalmente vi potranno essere testi al limite, ma questo appartiene ovviamente all'autonomia discrezionale e di valutazione dei Presidenti di Commissione e del Presidente del Senato.

prendiamo anche atto, però, della volontà di dedicare nei prossimi giorni, appena sarà possibile, una seduta della Giunta, per avere quindi un deliberato della medesima, su questa materia per mettere un punto fermo nel senso da lei stesso auspicato. Insisto invece sul punto che

dovendo discutere fra poco di emendamenti che sono chiaramente estranei all'oggetto del decreto e che, in virtù della prassi innovata ovvero del *decisum* della Giunta per il Regolamento che verrà, sarebbero oggi inammissibili, di ritirare gli emendamenti o comunque di trasformarli in ordini del giorno. Avremo numerosi altri provvedimenti nelle prossime settimane e mesi a cui eventualmente agganciare le norme, a partire dalla legge finanziaria, seppur di

«La 1a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.300, sul quale il parere è non ostativo, a condizione che l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto sia preceduta dall'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni». Conferenza Stato-Regioni». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo» ad eccezione delle proposte 3.0.4 e 3.0.7, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.0.3, 2.0.5, 3.2, 3.3, 3.6, 3.11, 3.0.5, nonché parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.2, 3.1, 3.4 e 3.0.9. Esprime poi parere di nulla osta sulla proposta 3.5 (testo 2) a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole: "pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 22,1 per l'anno 2009, si provvede", siano sostituite dalle altre: "si provvede nel limite massimo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 22,1 milioni per l'anno 2009,". Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti». (*Segue* AMATI, *segretario*). «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 (testo 2), 2.0.102, 3.0.8 (testo 3.0.3 (testo 2), 2.5, 1.0.4 e 3.5 (testo 2), nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.10, 3.0.4 (testo 2), 3.0.7 (testo 2) e 2.6 (testo 2). Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti».

qualche sfasatura che stavamo cercando di capire. Potete comprendere anche il lavoro che si sta facendo per portare in porto questo importante provvedimento. Per quanto

per i quali le rimodulazioni dell'elenco annuale dei lavori comporterà grosse difficoltà nella realizzazione delle opere. Infatti, l'incidenza delle varianti in corso d'opera si sente evidentemente di più nelle realtà dove questo numero di opere è limitato. D'altra parte, i Comuni con scadente progettualità (magari con un'unica opera da realizzare) potranno accedere direttamente al fondo governativo di 300 milioni di euro. Quindi, questi Comuni non risentiranno dell'aumento dei prezzi. Con questo emendamento, noi riteniamo utile far accedere al fondo governativo tutti i piccoli Comuni fino a 5000 abitanti.

ai tecnici comunali e, per la restante parte, al capitolo delle entrate del bilancio dello Stato. Chiaramente, ciò penalizza gravemente i Comuni, mettendoli nell'impossibilità di fatto di potere affidare

noi proponiamo di alzare l'importo dei lavori per i quali è ammessa la trattativa privata senza pubblicazione del bando di gara, poiché riteniamo che il vecchio importo di 100.000 euro sia attualmente una cifra assolutamente inadeguata

il terzo correttivo del codice dei contratti pubblici ha previsto all'articolo 32 la gara per le opere di urbanizzazione, realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nei casi di rilascio del permesso di costruire. del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede comunque l'espletamento di una gara, con invito rivolto ad almeno cinque concorrenti. Con questo emendamento, noi intendiamo escludere dalla gara le opere di urbanizzazione sotto soglia, lasciando disciplinare tali opere dalle norme che già disciplinano le convenzioni (in questo caso stipulata tra il richiedente il permesso di costruire e il Comune). Anche questa misura va nell'ottica del massimo snellimento di tutte le procedure che che determinano le condizioni per i piccoli Comuni di vedere realizzate le opere di urbanizzazione.

nell'ambito del quadro economico tra le somme disponibili per imprevisti o utilizzando il ribasso d'asta. Quando quelle risorse non fossero sufficienti o mancasse l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta, si determinano altri meccanismi. Noi proponiamo di garantire la copertura dei 300 milioni determinando un prelievo dalle risorse previste e disponibili nei programmi che finanziano la singola opera; in questo modo, si potrebbe anche superare il limite dei 300 milioni, perché potrebbero verificarsi situazioni che mettono in evidenza un divario ed un fabbisogno significativamente maggiore. Ove quelle risorse non fossero sufficienti, cioè il programma legge obiettivo o un programma regionale o un programma opere pubbliche comunale non avesse la necessaria disponibilità di risorse, noi proponiamo che a quel punto venga attivato un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, con oneri a carico dello Stato nel limite d'impegno fissato dalla legge finanziaria, per coprire il maggior fabbisogno derivante dall'incremento dei prezzi di cui ci stiamo occupando.

per evitare che si utilizzino, al solito, le risorse del FAS. Vorrei dire ai colleghi che sono intervenuti o a quelli che hanno registrato la discussione delle ultime sedute sulle questioni relative ai fondi FAS, che risultano di fatto depauperati attraverso il prelievo costante da quei capitoli, che la questione purtroppo non riguarda - devo dire -soltanto il Mezzogiorno d'Italia, perché provo già ad immaginare gli interventi e le preoccupazioni che emergeranno quando ci si renderà conto che i programmi operativi regionali delle Regioni del Centro-Nord non potranno partire perché risulterà insufficiente la dotazione regionale, dal momento che i profili finanziari di quei programmi operativi risultano cofinanziati con il FAS. questione, quindi, ha un impatto ben maggiore di quanto è emerso finora perché - figurarsi - del Mezzogiorno ci si può anche dimenticare, ci si può anche non preoccupare, provo ad immaginare quello che succederà quando ci si renderà conto che le scelte fin qui compiute determinano una paralisi nella utilizzazione delle risorse comunitarie. Per questo motivo, con l'emendamento 1.15 proponiamo una diversa copertura del necessario fabbisogno, superando anche la limitazione proposta dalla Commissione, assumendo il tetto dei 300 milioni di euro a garanzia delle imprese che hanno dovuto far fronte a costi imprevisti determinati da una modificazione non prevista e non prevedibile dei costi delle materie prime, come ripetutamente richiamato in questo provvedimento.

in omaggio ed in coerenza con quanto è stato dichiarato dal senatore Legnini. Ovviamente, questo vuole essere implicitamente anche un invito ai colleghi a ritirare gli emendamenti che esulano totalmente dai temi oggetto del provvedimento. Credo sia importante partire dall'esempio;

Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 ha il fine di tutelare il comparto del commercio di materiali edili, costituito in maggioranza da piccole e medie imprese. Questo comparto registra situazioni di sofferenza nella riscossione dei pagamenti in misura notevole e superiore rispetto a quella di altri settori commerciali. Ciò è dovuto in larga misura alla circostanza che le imprese di costruzione, ed edili in genere, tendono a differire pagamenti dovuti ai propri fornitori di materiale all'avvenuto incasso dei corrispettivi per l'appalto o per le prestazioni d'opera. Si rende, pertanto, indispensabile questa previsione normativa di rimedi più consoni al normale andamento delle pratiche negoziali di impresa,

del commercio nel settore dell'edilizia, che sta soffrendo particolarmente nella riscossione dei pagamenti rispetto ad altri settori. Ciò è dovuto alla prassi, ormai invalsa, tra le imprese di costruzione a differire i pagamenti nel momento in cui ricevono i pagamenti dall'appaltante. Spesso questo accade anche con maggiore ritardo, ovvero anche successivamente alla

un problema noto a tutti, vale a dire i ritardi di pagamento della pubblica amministrazione nei confronti di aziende, di soggetti diversi, problema che ormai sta raggiungendo dimensioni non più tollerabili in un Paese civile. Stiamo raggiungendo in alcune Regioni punte di 400 giorni di ritardato pagamento, e comunque la media nazionale tende ad essere di 300 giorni. Il complesso delle risorse che hanno questo ritardato pagamento sta raggiungendo i 70 miliardi euro. Resta evidente a tutti noi, signor Presidente, che una situazione di questo genere compromette fortemente il funzionamento e, a mio avviso, anche la sopravvivenza di molte imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni. Questo, infatti, si sta aggiungendo ad un situazione di estrema difficoltà di accesso al credito,

a soluzione questo problema. Da una parte si propone la compensazione fiscale, invertendo quindi un principio oggi in atto, vale a dire quello secondo cui l'impresa che è debitrice fiscalmente nei confronti dello Stato si vede bloccare i pagamenti, ma nel contempo l'impresa creditrice nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve comunque continuare a pagare allo Stato ciò che deve. Noi chiediamo che deve. Noi chiediamo che ci sia compensazione rispetto a questo dato. In secondo luogo, laddove non ci sia la possibilità di compensare, si propone un altro tipo di soluzione, vale a dire la possibilità per la pubblica amministrazione di certificare

il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, un sistema che consenta di avere il credito certificato della piccola e media impresa come strumento per avere scontato in banca - che oggi inizia

non sia essere superiore a quello Euribor. Contestualmente si prevede anche l'intervento della Cassa depositi e prestiti, oltre che di Confidi,

quelle realtà e quei Comuni che abbiano una situazione di tardato pagamento legata al patto di stabilità e non ad inefficienze di altra natura. La proposta è articolata, sostenibile tende a dare una soluzione a un problema che sta diventando di assoluta criticità, attraverso la modalità che ho illustrato e che risponde a diverse tipologie di motivazione di tardato pagamento.

non vengono attuate le disposizioni di direttiva comunitaria che prevede, rispetto ai tardati pagamenti ulteriori ai 30 giorni, l'applicazione di tassi d'interesse almeno di sette punti superiori ai tassi della BCE. Ciò non avviene; anzi, quando le imprese vanno in giudizio, normalmente si vedono poi costrette a compensare anche le spese di giudizio. Anche questo si aggiunge alle loro difficoltà.

il quale si auspica la compensazione tra debiti e crediti per i fornitori dello Stato. All'epoca trovai nella maggioranza molte persone d'accordo su questo

molto bene illustrato dalla collega Leddi, riguarda un tema molto delicato ed abbastanza rilevante. Ne chiedo la trasformazione in un ordine del giorno

l'emendamento 1.0.400 e di trasformarlo in un ordine del giorno.

sono decisioni che si possono prendere *ex* articolo 100 del Regolamento, perché è stata una decisione abbastanza discussa. Pertanto, la prego, signor Presidente,

Credo che ci siano le condizioni per poterlo riesaminare, però naturalmente è una decisione che va presa in sede di Commissione, per cui chiedo cortesemente al relatore di accantonarlo, di esaminarlo per ultimo, e lo riconsidereremo in Commissione alla fine dei lavori.

naturalmente noi parteciperemo ai lavori della Commissione stessa e formuleremo nuovamente il nostro parere. La mia opinione è comunque

di proventi che l'ANAS percepisce in ragione di un aumento dei canoni di concessione alle concessionarie, che dovevano essere rigorosamente impiegati (tra l'altro la questione è oggetto di una mia

da par suo, ha riportato le cifre non impiegate negli esercizi futuri impegnandosi in Commissione sostanzialmente ad assolvere a questa funzione. Noi chiaramente ne chiederemo in finanziaria la destinazione ad altre autorità di vigilanza che non hanno potuto

che è un argomento già affrontato in Commissione. Si tratta di risorse di una certa consistenza che possono essere utili anche ai fini di questo provvedimento. Pertanto, credo che l'emendamento in esame vada mantenuto per agevolare l'attività dell'ente. Peraltro, si tratta di una regolazione che va fatta più in generale nel contratto di servizio tra l'ANAS Spa e e l'azionista. Quindi, in quella sede verrà meglio affrontato il tema dell'utilizzo di tali risorse provenienti dai ticket autostradali esclusivamente o meno

diverse dai trasferimenti di tipo ordinario non vedo come si possa farlo. Credo pertanto che questa norma vada mantenuta.

ANAS, il senatore Marco Filippi le ha chiesto di invitare i proponenti a ritirarlo. Infatti, se fossero applicate le norme che questa mattina il Presidente, in accoglimento delle nostre istanze, ha detto che saranno applicate nel prossimo futuro, esso sarebbe stato dichiarato inammissibile.

fate uno sforzo, come stiamo facendo noi, e ritirate questi emendamenti, che evidentemente sono estranei all'oggetto della discussione. Senatore Legnini, capisco la solidità del ragionamento, ma non posso che confermare la risposta che già oggi il presidente Schifani ha dato sull'argomento in questione. Ovviamente resta alla decisione dei Gruppi la possibilità di regolarsi come meglio credono.

di fatto dà soluzione ad un problema reale e oggettivo che il nostro Gruppo condivide pienamente. Siamo consapevoli dell'impossibilità attuale di inserirlo in una norma.

alle imprese e alle famiglie, in arrivo, si tenga conto di questa che può essere un'ottima soluzione, oltretutto a costo zero,

sia possibile largamente condividere nel Senato tra maggioranza e opposizione. In questo momento noi tutti lamentiamo che le imprese piccole, piccolissime, medie e grandi subiscano, anche se si dice contrario, il contingentamento del credito da parte degli istituti di credito che, per loro ragioni e difficoltà, tendono a - se vogliamo usare una espressione eufemistica - lesinare il credito nei confronti delle imprese.

consentiremmo alle imprese di avere un alleviamento del peso derivante dal contingentamento del credito per questa via. È per questo che, a mio giudizio, nel provvedimento un emendamento di questo tipo - questo sì avrebbe carattere d'urgenza e servirebbe ad alleviare le condizioni di gravissima difficoltà in cui versano le imprese e mi auguro che

nelle diverse sedi a favore delle piccole imprese, non si facesse questa che è la principale misura per aiutare le imprese di fronte alle difficoltà della crisi finanziaria che intanto potremo prendere nell'immediato. *(Applausi dal

la parte che ovviamente interessa la Commissione bilancio è la seconda, quella inerente alle coperture, mentre la prima parte è di natura procedimentale. Poiché si sta tentando di recuperare la prima parte sul testo che diventerebbe vigente, quello del Governo,

mi collego al ragionamento che veniva testé fatto dal relatore. L'emendamento 2.100 verrà ritirato nel momento in cui il relatore

senatore Zanetta

al Presidente della Commissione difesa: era certamente un argomento da affrontare in quella sede. Quindi, il ritiro è più che giustificato anche per tutto il dibattito che su questo tema si è svolto in Aula.

a firma dei colleghi Benedetti Valentini e Bornacin, tende a risolvere un problema che si trascina da anni e che penalizza fortemente le imprese che fabbricano semirimorchi destinati all'esportazione. Infatti, in virtù di una una soppressione, disposta a mezzo di una circolare, della possibilità di trasportare veicoli su veicoli si è determinata una riduzione di competitività, con maggiori costi per il trasporto, in danno delle imprese italiane ed a vantaggio dei concorrenti europei. Si tratta di una norma di semplice fattura, che non comporta oneri e che è attinente all'oggetto del decreto, trattandosi

abbattere i costi di trasporto, contribuendo peraltro anche a non accrescere l'inquinamento. È infatti evidente che se due o tre veicoli devono viaggiare distintamente producono maggiori consumi e maggiore inquinamento che se viaggiassero caricati l'uno sull'altro, come avveniva fino al 2003; poi, nel 2004, una circolare ministeriale, credo erroneamente, ne dispose la soppressione. Signor Presidente, consento con tutte le considerazioni che ha svolto ora il senatore Legnini.

dubbi favori al settore industriale della mobilità, più o meno trasparenti e accettabili. In questo caso, senza spese

come facciamo ad esaminare gli altri emendamenti, sussistendo la possibilità che l'intero articolo venga sostituito? Francamente, io non comprendo il senso di una procedura di questo tipo: 2.200 non si accantona o, se si accantona, bisogna accantonare molti altri emendamenti. In ogni caso, va valutata bene la conseguenza della decisione di accantonamento.

Per organizzare un evento di questa portata, il Governo ha ritenuto legittimamente, e direi doverosamente, non solo di attuare la programmazione ordinaria per le spese necessarie alla realizzazione di questo evento mondiale, ma anche di esprimersi con i contatti canonici tra Stato e Regioni e con le deliberazioni di provvedimenti, le ordinanze della Protezione civile. L'emendamento si è reso necessario per mettere a punto fondamentalmente due aspetti: il primo relativo alle riposizionamento di un terzo delle spese complessive a carico del FAS interregionale. Nel testo presente in questo decreto e difformemente da quanto concordato dal Presidente del Consiglio con le Regioni e da quanto espresso dallo stesso Presidente del Consiglio con una propria ordinanza, circa un terzo, ammontante all'incirca a 100 milioni di euro, verrebbe spostato dal FAS interregionale al FAS regionale. Quindi, un evento che viene ospitato in Sardegna, con la soddisfazione di tutti, di fatto verrebbe a costare, in maniera noi riteniamo impropria e comunque non dovuta, alla disponibilità del Fondo relativo, nello specifico, della Regione sarda. Si chiede anche, signor Presidente, illustri colleghi, che le opere definite accessorie, ma non per questo meno importanti per garantire il funzionamento delle delle manifestazioni del G8, possano essere attivate con la dovuta speditezza. Ho il piacere di avere di fronte, in questo momento, colleghi autorevolissimi della maggioranza che conoscono quanto me e forse meglio di me i problemi di cui sto parlando; loro sanno, ad esempio, che se questo testo del decreto rimanesse com'è, se cioè questo emendamento non venisse accolto, si interromperebbe, nonostante un'esplicita ordinanza del Presidente del Consiglio ed una altrettanto esplicita affermazione del sottosegretario Bertolaso resa qualche giorno fa alla Camera, la fase di

in uno spirito e con un atteggiamento assolutamente *bipartisan*, senza che ci si accapigli per sventolare più in alto degli altri le bandierine, mi appello a lei, signor Presidente, ed ai colleghi della maggioranza per rendere possibile un avvenimento di straordinaria importanza, qual è appunto il G8, grazie al conforto ed al sostegno di iniziative e di determinazioni poste a carico dell'intero Paese e non a carico della sola Regione Sardegna, favorendo quella celerità delle decisioni senza la quale gli impegni assunti formalmente dal Capo del Governo non potrebbero realizzarsi.

una questione essenziale che è stata adombrata dal collega Scanu. Ci troviamo di fronte ad una scelta di politica estera, e soprattutto della sicurezza, in virtù della quale la Maddalena viene scelta come sede del G8 per l'anno È davvero singolare che i costi di un evento di politica estera, determinato da ragioni di sicurezza, vengano posti a carico della Regione che ospita il G8. Questo vale per il caso in questione e ovviamente deve valere per tutti i casi; quindi, chiederei veramente ai colleghi di considerare con un minimo di distacco e di serenità questo dato di fatto.

cerca di chiarire un concetto fondamentale, ovvero che il beneficio della sospensione, previsto dall'articolo 3, in particolare modo la modalità attraverso la quale vengono restituiti i tributi e i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, che è ridotta al 40 per cento in 120 rate mensili, si estende anche al settore pubblico. Si conferma perciò che tutti coloro che hanno fruito del beneficio della sospensione

recita testualmente: «La legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile». In ordine a ciò sta accedendo che INPS e INPDAP,

ritengono che debbano essere esclusi dalle disposizioni di ammissione alla restituzione in forma ridotta al 40 per cento in 120 rate mensili i datori di lavoro e i lavoratori pubblici. pubblici. Conseguentemente, con diversi provvedimenti si stanno adoperando per richiedere la restituzione dei contributi a dipendenti e datori di lavoro pubblici, con modalità diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 3 del disegno di legge

Marche ed Umbria, che hanno subito gli effetti del sisma del 1997.

di concretezza a un territorio che, come accennava la senatrice Fioroni, ha subito il sisma del 1997 e che ora si trova a combattere con una crisi economica che sta minando tante piccole e medie aziende, e quindi tante famiglie,

dei tributi e dei contributi, che era stata portata al 20 dicembre 2008. Avevamo tutto il tempo per legiferare in materia. Oggi invece non c'è più tempo;

del G8 vengano gestiti con ordinanze della protezione civile. Occorre che questa legge venga rivista, perché in essa debbono essere fissati i diritti della gente. Non è possibile che i deboli del Molise vengano trattati in maniera diversa da quelli di altre Regioni. Tutta l'Italia dovrebbe avere le stesse regole per ciò che riguarda la sospensione e la restituzione. Non faccio il mendicante, né l'accattone, ma chiedo diritti.

30 ordinanze diverse, l'una contro l'altra e stanno avvenendo delle vere e proprie tragedie nel nostro Molise.

Spesso sono stato accolto dal sorriso ironico. Oggi, invece, reclamo diritti e poiché tra pochi giorni vi sarà una cerimonia nel mio Paese che vedrà presente il Presidente del Consiglio, vorremmo accoglierlo bene, come si deve accogliere un amico, un rappresentante massimo delle nostre istituzioni, e non vorremmo ricorrere alla stampa per fare determinate cose.

tono e di essermi rivolto in modo duro. Ho sempre ringraziato tutti per la comprensione, ma oggi - ripeto - non posso più farlo, perché siamo veramente in uno Stato di non diritto per la popolazione della mia Regione o di quella piccola parte della mia Regione.

in Sardegna si verificavano eventi alluvionali molto gravi che hanno portato alla morte di cinque persone e danni per molte decine di milioni di euro.

preallocazione rispetto alla riprogrammazione che in queste ore il Governo sta discutendo con le Regioni e che nella giornata di domani sarà oggetto della discussione e della decisione del CIPE.

se le misure di agevolazione si estendono al settore pubblico e soprattutto ad invitare gli istituti INPS e INPDAP a emanare atti in cui informano gli enti pubblici delle Regioni Marche e Umbria circa l'estendibilità di queste misure anche al settore pubblico, nonché a quello assicurativo e bancario.

stiamo prendendo, tutti assieme i Paesi d'Europa, delle decisioni in ordine alla possibilità di reperire risorse per lo sviluppo che sicuramente terranno conto dell'opportunità di per cui sono stati istituiti, cioè per attenuare le differenze, a valle di questo processo. Già la manovra finanziaria che il Governo sta predisponendo

Signora Presidente, mi rendo conto della possibile irritualità di quanto sto per affermare e pertanto preliminarmente mi appello alla sua cortesia. Anche alla luce delle esplicite e apprezzate dichiarazioni rese poco fa dal collega Pisanu, in luogo di un'approvazione di questo emendamento, rispetto al quale il collega relatore ha manifestato ancora delle perplessità, ne vorrei in subordine chiedere

si riunirà per determinare la cosiddetta preallocazione dei fondi FAS, il che significa che gli auspici espressi dal relatore verrebbero fortemente resi più consistenti se già dalla giornata odierna il Senato si pronunciasse in questi termini, orientando in maniera sensibile il lavoro che domani il CIPE dovrà sviluppare. Quindi, con il suo consenso, signora

vorrei chiarire che né la maggioranza né il Governo potranno avere la coscienza a posto in merito ai danni che stanno facendo non approvando quegli emendamenti che davano dignità alle nostre terre. La verità è che voi, in questo momento, vi assumete una grande responsabilità rispetto alla vicenda dei FAS, perché non è assolutamente vero, caro collega Cicolani, che l'Europa ci aiuterà. Sono Sono tutte le bugie che ancora una volta stanno emergendo rispetto alla vostra politica che arrecherà danni nei territori di cui stiamo parlando. Presidente, al di sopra di qualunque senso di appartenenza, che ritengo di aver sempre professato a testa alta e mi auguro con onestà intellettuale, sento di dovermi comunque dichiarare soddisfatto

di un senatore che appartiene al Partito Democratico, il quale vorrà - se lo riterrà - esprimere le proprie argomentazioni politiche senza accavallarle,

per favore!

in assenza di una normativa nessuno sa come comportarsi, eccetto gli enti previdenziali, che naturalmente già stanno richiedendo i tributi e i contributi ai cittadini molisani. Inoltre, sono convinto che i cittadini italiani, di fronte allo stesso problema, dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Chiediamo che per il Molise siano adottati gli stessi provvedimenti proposti in questo disegno di legge per l'Umbria e per le Marche.

degli interventi finanziari per portare a termine questa benedetta ricostruzione (ormai abbiamo superato il decennale dagli eventi sismici). Tuttavia al momento

delle seconde abitazioni o delle situazioni particolari che è ancora ben lungi dall'essere risolta. Pregherei pertanto la collega Fioroni e gli altri firmatari di evitare una bocciatura, che sarebbe contraria agli intendimenti dell'Assemblea e credo anche del Governo, oltre che nostri,

a CAI, ma che per tale via stanno determinando uno stravolgimento delle disposizioni in materia di procedure concorsuali e, in questo specifico caso, lo stravolgimento di una norma estremamente consolidata posta a presidio dei diritti dei lavoratori,

vogliono eliminare totalmente le garanzie previste per i lavoratori dall'articolo 2112 del codice civile, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda

- che, nel caso in cui si proceda alla cessione dell'azienda o del ramo di azienda di una grande impresa in crisi, i rapporti di lavoro relativi a quella porzione di azienda si trasmettono automaticamente alla cessionaria dell'azienda stessa e i lavoratori mantengono tutti i diritti pregressi, oltre ad

di Alitalia e AirOne a CAI. Si tratterebbe cioè di determinare una separazione tra la vecchia e la nuova gestione. Non c'entra assolutamente nulla, signora Presidente. A me non risulta (ma credo non risulti a nessuno) che l'Europa ci chieda di violentare e di abrogare i diritti dei lavoratori delle aziende in crisi. Non c'entra nulla!

in tutte le aziende in crisi i lavoratori dovranno recarsi con il cappello in mano presso l'azienda cessionaria per ottenere il ripristino del rapporto di lavoro che, altrimenti, non è in alcun modo tutelato. È un fatto molto grave, signora Presidente, anche perché questa disposizione applicata nel futuro determinerà le condizioni per una elusione dei diritti dei lavoratori, come determinerà

Fatelo! Ve ne assumete la responsabilità! Scriviamo però in questa norma, signora Presidente, signori del Governo (vedo presente anche il ministro Matteoli), signor relatore, che essa si applica solo ad Alitalia

ripeto, sopprimendo di fatto anche il diritto di credito dei lavoratori nei confronti di Alitalia che non sarà in alcun modo soddisfatto. Ripensateci. Avete proceduto all'accantonamento di diverse norme, peraltro non accogliendo le indicazioni venute dal dibattito che si è svolto ieri e oggi sulla improponibilità e sull'inammissibilità

rischia di essere vano per Alitalia e di valere solo per le altre aziende. Infatti, questa mattina i giornali riportano che la cessione del ramo di azienda di Alitalia a CAI si perfezionerà domani o dopodomani, comunque nei prossimi giorni;

la particolare forma di rapporto scelta tra gli attuali proprietari di Alitalia, Alitalia e CAI cozza su di un punto con la normativa comunitaria. Infatti quella che per la normativa comunitaria si profila - esplicitamente, a mio giudizio - come cessione di un ramo di azienda noi non non la stiamo qualificando come tale. Non sto dando un giudizio, sto semplicemente descrivendo la situazione. Questo potrebbe determinare in sede comunitaria una procedura di infrazione da cui lo Stato italiano, a mio giudizio, uscirebbe certamente soccombente - per avere effettuato secondo regole non corrispondenti a quelle comunitarie la cessione di un ramo d'azienda.

Senonché, le conseguenze sono paradossali rispetto al movente dell'emendamento: approvando una norma che vale *erga omnes*, praticamente eliminiamo dal nostro ordinamento la figura della cessione del ramo d'azienda, del tutto coerente

studiamo una norma che ci consenta di non avere questo problema, ma non approviamo una norma di questo tipo *erga omnes*, che potrebbe avere gravi conseguenze sociali. In una situazione in cui si stanno moltiplicando le crisi dei grandi gruppi industriali, che potrebbero dar luogo ad amministrazione straordinaria con successiva cessione di rami d'azienda, potremmo stare decidendo, senza saperlo, di introdurre nel nostro ordinamento una cessione di ramo d'azienda che avviene in assenza di tutele per i lavoratori del ramo del ramo d'azienda stesso. Francamente non riesco a pensare che la maggioranza voglia assumere una iniziativa di questo tipo e quindi la invito caldamente a ripensare il testo di questo emendamento. *(Applausi

astenere dall'ennesimo pasticcio che stiamo facendo in questa vicenda Alitalia. Vorrei ricordare che esiste una direttiva europea che definisce e regola il trasferimento d'azienda e rispetto alla quale il legislatore nazionale non ha la potestà di stabilire che cosa è trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda e cosa non lo è. L'operazione che stiamo facendo è sicuramente destinata non soltanto ad essere cassata dalla Corte di giustizia, ma ad esporre lo Stato italiano ad una sanzione per violazione di quella direttiva. In ogni caso non solo non salverà l'operazione CAI-Alitalia dalla censura comunitaria, ma creerà un ulteriore ostacolo alla nascita della nuova compagnia. Stiamo attenti a non aggravare i danni che abbiamo già fatto e che si stanno verificando in questa pasticciatissima vicenda.

ci troviamo di fronte a licenziamenti, a chiusure, a cessioni di rami d'azienda in molti settori produttivi di questo Paese. di colpire centinaia di migliaia di lavoratori, i loro diritti e le loro condizioni economiche. È un errore gravissimo, che poi sull'insieme del Paese. Ripensateci su a questo punto, perché è una prospettiva veramente drammatica. Volete farlo per l'Alitalia? Fatelo, anche se non serve a niente. Ma non colpite tanti lavoratori e tante lavoratrici, soprattutto dei settori più deboli!

di alcuni aspetti di questa normativa quando arrivò in Commissione, e allora c'era un tentativo, da parte della maggioranza, di distinguere e di ridurre l'applicabilità delle norme di tutela in questo caso. Adesso, invece di correggerci, stiamo rincarando la dose, nel senso che si vuole eliminare del tutto l'applicazione di una norma fondamentale che si richiama ad una direttiva europea.

tra cui questo - di cambiamenti di assetti azionari e di trasferimenti di realtà imprenditoriali. Se non cambiamo o ritiriamo questa norma rischiamo di andare esattamente contro una tendenza generale dell'Europa, ma anche di altri Paesi, e veramente contro le elementari necessità di giustizia sociale. A questo anch'io mi appello e, comunque sia, una norma del genere verrebbe sicuramente condannata dalla Corte di giustizia, quindi su questo non possiamo transigere.

della nostra Commissione, alcuni aspetti sono stati analizzati e posti all'attenzione del Governo, il quale ritiene però che questa posizione debba essere confermata anche per profili di costituzionalità.

un'azienda che produce acciaio, la Thyssenkrupp, com'è stato a lungo discusso, questo emendamento, se approvato, metterebbe in pericolo tutte le produzioni strategiche ad alto assorbimento di energia (mi riferisco in particolare al settore dell'alluminio), con gravi ricadute economiche e occupazionali per il Paese, ma anche per i territori dove queste produzioni industriali sono insediate. Mi riferisco in modo ancora più specifico a Porto Marghera e alla Sardegna. se ce n'è fosse bisogno, in piena crisi economica si colpisce un comparto, appesantendo ed aggravando, con una certa superficialità e improvvisazione, la già difficile condizione della nostra politica industriale. Si dice che questo ci viene richiesto dall'Europa, eppure tutti i Paesi europei sono alle prese con l'applicazione di queste norme comunitarie, ma nessuno sta pensando di dismettere un comparto industriale con tale improvvisazione e senza una chiara strategia produttiva in questi settori. Il riposizionamento del settore dell'alluminio è una questione strategica anche dal punto di vista delle produzioni e prima di dismettere un settore come questo bisognerebbe attrezzarsi con un piano di ristrutturazione industriale che consentisse di tenere conto sia della necessità di produzione per l'autonomia del Paese sia delle ricadute occupazionali ed economiche che si prefigurano. Credo sarebbe utile evitare di fare ancora del male al nostro Paese nel momento di grave crisi generale che sta attraversando l'economia.

una riflessione, ho avuto l'impressione, nel corso del dibattito in Aula, che vi siano altri emendamenti da riesaminare. La Commissione bilancio non si sottrae al compito di un riesame, ma questa prassi è al limite dell'irritualità. La revisione di un nostro parere è un fatto assolutamente eccezionale che, se giustificato dal dibattito avvenuto in Commissione o da quello in Aula o da una posizione del Governo o del relatore, risulta comprensibile e la Commissione bilancio lo fa volentieri.

di rivedere il nostro parere qualora fosse effettivamente possibile, avendo però ben chiaro che si tratta di una soluzione assolutamente eccezionale e che il nostro parere riguarderà solo gli effetti finanziari, rimanendo le questioni di merito deferite

i senatori della Commissione agricoltura sono sicuramente edotti in materia - che durante la notte è stato raggiunto a Bruxelles un importante accordo in sede di revisione della Politica agricola comune, il cosiddetto *Health check*. Credo che questo possa essere giudicato un accordo fortemente migliorativo rispetto alla proposta iniziale della commissaria Fischer Boel; un accordo positivo il quale l'Italia ha svolto un ruolo veramente importante, propulsivo (di questo va dato atto) grazie all'azione decisa, importante e determinata del ministro dell'agricoltura Zaia, a cui va il nostro ringraziamento *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP)* e con la partecipazione del Presidente del Consiglio, che personalmente è intervenuto scrivendo una lettera al presidente Barroso. Quindi, è un grande successo per l'agricoltura italiana, che risponde anche al malessere che vi è in questo momento nelle campagne.

di una notevole recrudescenza, perché le trattative negli ultimi tempi hanno portato alla situazione disastrosa che l'agricoltura italiana sta vivendo in questo periodo. Speriamo sia - come effettivamente è - l'inizio di una nuova era per l'agricoltura italiana.